Dichiaro aperta la votazione.

Presidente, prima di iniziare l'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria, vorrei comunicare all'Assemblea che il Gruppo di Alleanza Nazionale ritira un certo numero di emendamenti.

ma oggi intervengo all'inizio della seduta, e mi pare che lo spazio necessario e sufficiente ci possa essere,

dell'Aula uno dei problemi più inquietanti di fronte ai quali a me pare che non solo la società italiana, ma tutta la politica si dichiari come impotente (lo faccio a seguito dell'ennesimo episodio doloroso): il problema della violenza che si manifesta nei ragazzi, nei preadolescenti e negli adolescenti verso i loro coetanei, loro coetanei, e il fenomeno che chiamiamo in modo eufemistico bullismo (non abbiamo altre parole, quasi a voler esorcizzare la verità), cioè la mancanza di rispetto per l'altro e l'aggressione dell'altro. Lunedì scorso a Roma un ragazzo di quattordici anni italo-marocchino (non era il primo e temo che non sarà l'ultimo) è stato preso a pugni e a catenate dai suoi coetanei.

Talvolta le molestie covano a lungo e poi esplodono. Ragazzi derisi e umiliati si sono suicidati. Signor Presidente, colleghi dell'Aula, mi pare che non dobbiamo spendere altre parole. C'è un'emergenza educativa nel nostro Paese. È un'emergenza culturale e civile: vi è una *escalation* inquietante. L'emergenza più seria è questa: la paura, già presente nella società, è entrata nella scuola, la paura e la difesa da chi è diverso, mentre la scuola è per eccellenza il luogo dell'incontro, della scoperta dell'altro e dello scambio. Siamo nell'imminenza di elezioni studentesche. Vi sono liste con riferimenti al fascismo e alla xenofobia. Ieri il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto ai capi di istituto più vigilanza. L'ha chiesta anche al Ministro dell'interno.

7a Commissione del Senato, all'unanimità, ha presentato per l'Aula una risoluzione sull'insegnamento della Costituzione italiana nelle scuole del nostro Paese. Siamo nell'imminenza del passaggio dei sessanta anni dalla scrittura della Costituzione e dalla sua promulgazione. Le chiedo, se è possibile, nelle prossime settimane, di dare voce

In secondo luogo, da anni in Italia ogni giorno centinaia di ragazzi italiani vengono derisi, insultati e picchiati da coetanei stranieri e nessuno dell'Unione si è sentito di intervenire in quest'Aula. *(Applausi

Presidente, in questi giorni abbiamo letto sui giornali e ascoltato trasmissioni televisive cui autorevoli esponenti del Governo hanno dichiarato che il voto di fiducia sulla finanziaria non ci sarebbe stato se l'opposizione non avesse praticato l'ostruzionismo. *In primis*, il ministro Chiti ha dichiarato però che i circa 550 emendamenti presentati dall'opposizione erano un numero enorme. Vorrei fare presente all'Aula, che lo sa sicuramente meglio di me, che dal 2000 ad oggi mai erano stati presentati dalle opposizioni così pochi emendamenti come in questa circostanza.

Abbiamo sentito anche in quest'Aula, credo per la nota ignoranza costituzionale da parte di un Ministro della Repubblica, che non si esclude la fiducia sulla finanziaria. Non vi sarebbe alcuna giustificazione, perché abbiamo detto fino alla noia, ed è bene che i colleghi della maggioranza lo sentano, che garantiamo comunque il rispetto del termine del 14 novembre. però, che grazie alla cortesia di tutti i colleghi senatori dell'UDC il Gruppo ha dimezzato i propri emendamenti. Poiché questa maggioranza non consente di parlare neanche per illustrare il ritiro degli emendamenti,

arrivati al momento della verità per tutti. È opportuno che questo momento della verità giunga attraverso un percorso fisiologico

il significato preciso che vogliamo dare all'ulteriore sforzo che abbiamo fatto. Ringrazio i colleghi del mio Gruppo che hanno accettato il sacrificio di ritirare qualche emendamento. Consegneremo quanto prima alla Presidenza Signor Presidente, non ripeto le motivazioni di carattere politico, perché già esposte dai colleghi che mi hanno preceduto. Noi della Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano non abbiamo presentato sin dal principio e per gli stessi motivi un gran numero di emendamenti. In tutto erano una ventina e, di essi, ritiriamo il 13.0.1, il 14.11 e il 38.2.

saranno votati nella forma stampata nel fascicolo con l'intesa che, in caso di approvazione, gli articoli aggiuntivi saranno soggetti a coordinamento finale. Comunico che l'emendamento 3.804 è improponibile ai sensi dell'articolo 128, commi 3 e 4, del Regolamento in quanto non risulta respinto in 5a Commissione né si trova in correlazione con le modifiche proposte dalla Commissione stessa. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.300, 3.804 (limitatamente al comma 2-*nonies*), 7-*ter.* 801 e 49-*ter.*800. Il parere non è ostativo sulle restanti proposte emendative».

ma non ha detto perché, per la prima volta nella storia della Repubblica, l'Assemblea è chiamata a votare un emendamento privo della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. La richiesta che ripropongo è la seguente: il Ministro dell'economia spieghi perché in quell'unico emendamento non

della pseudoriduzione di tasse che l'anno scorso è stata sbandierata. Come ad ogni ciclo delle stagioni, ad ogni primavera arriva qualcuno del centro-sinistra che dice che ridurrà le tasse. Quest'anno invece ci siamo accorti che anche le tasse dei lavoratori dipendenti sono importanti e vogliono ridurle d'accordo con il sindacato. Da tempo la Lega diceva che si potevano detassare gli aumenti

di quanto ho avuto modo di affermare ieri in sede di discussione generale, quella cioè di cercare di rovesciare la tendenza che ci sembra propria di questo Governo del tassa e spendi, spendi, fissando, quindi, un paletto preciso rispetto alla ipotesi che si verifichino entrate maggiori di quelle che sono state preventivate dal Governo,

ridurre innanzitutto il *deficit* e successivamente la pressione fiscale. Abbiamo preso per buona la cifra indicata dal Governo nell'allegato 8 alla finanziaria che aveva presentato, cioè 426.708 milioni al netto delle regolazioni contabili e debitorie; cifra che troviamo poi confermata anche nelle tabelle allegate al testo licenziato dalla Commissione. Conseguentemente, partendo da questo dato, che le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nello stesso esercizio vanno prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal dal DPEF (ed in questo non modifichiamo la previsione contenuta nel testo della Commissione). siano eccedenti rispetto a tali obiettivi prevediamo invece una destinazione diversa da quella decisa dalla Commissione cioè che debba essere istituito un apposito fondo, denominato fondo per il giusto indennizzo fiscale, da destinare, con successivi provvedimenti, esclusivamente al taglio lineare dell'IRPEF e dell'IRES, non ad una riduzione selezionata come quella che prevede la Commissione. Questo ci sembra rispondere ad una logica, secondo noi, fondamentale, quella di indicare una volontà precisa da parte del Parlamento di ridurre la pressione fiscale qualora dovessero giungere ulteriori entrate, dopo che queste sono state destinate alla riduzione del disavanzo, e porre, ripeto, un paletto al tentativo di spendere questi quattrini in modo indiscriminato. Questa è la logica del mio emendamento che raccomando al voto dell'Assemblea. Signor Presidente, i due emendamenti insistono sull'ormai noto comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria,

di optare, per l'eventuale extragettito del 2008 derivante dalla lotta all'evasione avente carattere strutturale, quindi permanente, di destinare eventualmente, con apposito provvedimento nel corso del 2008, queste risorse alla riduzione della pressione fiscale su tutti i lavoratori dipendenti. La Commissione che un intervento sugli autonomi (e qui motivo il mio parere contrario all'emendamento 1.800) sia stato già effettuato con il testo della legge finanziaria. Ricordo ai colleghi Del Pennino e Polledri e ai colleghi dell'opposizione che la misura che riguarda le imprese cosiddette marginali, con fatturato sotto i 30.000 euro, è senza precedenti, è la più grande semplificazione, il più grande sostegno alle piccole e piccolissime iniziative imprenditoriali

in corso di anno approvato, dovrà partire da tali fasce) è finalizzato ad introdurre come beneficiari dell'eventuale riduzione della pressione fiscale anche gli autonomi. Ripeto, la riduzione della pressione fiscale per gli autonomi già è prevista nella legge finanziaria; si può opinare sulla congruità e sulle modalità ma già esiste ed esiste anche nella riforma IRES, laddove si consente ai soggetti piccole imprese, persone fisiche e soci di società di persone di optare per la più favorevole aliquota fissa del 27,5 per cento, a condizione che non prelevino gli utili dall'impresa. Quindi, del tutto serenamente e coerentemente con il deliberato della Commissione, esprimo parere contrario ad entrambi gli emendamenti. SARTOR,

Signor Presidente, noi voteremo convintamente a favore degli emendamenti 1.2 e 1.800, nella consapevolezza che l'operazione fatta dalla maggioranza

e non ad un'altra che ha gli stessi problemi? Perché ai pensionati no? I pensionati al minimo stanno meglio dei lavoratori dipendenti? Naturalmente non è credibile. L'unica cosa credibile è che questa maggioranza fa dell'invidia sociale un meccanismo di Governo, cerca di aizzare gli animi gli uni contro gli altri. Questo è l'unico ragionamento politico ed economico che sta dietro alla proposta di redistribuire solo ai dipendenti e non ai disoccupati, non ai pensionati, non ai poveri. È una cosa assolutamente incomprensibile. Per questo motivo voteremo convintamente per l'espunzione di questa norma aberrante dal punto di vista logico, intellettuale e morale dalla legge finanziaria.

sulla portata politica ed economica della norma che è stata approvata in Commissione. Ho già detto nel corso della discussione generale che la questione della discriminazione che viene sollevata, in particolare dall'emendamento 1.800, non si pone, perché nel nostro sistema fiscale pacificamente e da anni è previsto che la detrazione per le spese di produzione del reddito sia diversa a seconda della attività del soggetto contribuente; questo è un caposaldo discutibile quanto si vuole, ma è un caposaldo del sistema

una norma di tipo fiscale che, affrontando il tema dell'aumento o della diminuzione, in ogni caso di un intervento sulla detrazione per spese di produzione del reddito, ipotizzi di agire tenendo conto della distinzione che è già fatta dal sistema a regime tra lavoratori dipendenti e pensionati da una parte e lavoratori autonomi dall'altra, non è questione che si pone o che si può porre, a mio parere, fondatamente nella chiave di chi denuncia una discriminazione. Se si passa da questo punto di principio al merito, poi, si vede che l'intervento che noi proponiamo, che è stato approvato dalla Commissione, Commissione, è volto ad affrontare quella questione salariale nel nostro Paese che, a mio giudizio giustamente e finalmente, è stata posta al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica italiana ormai non solo dagli interventi dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, delle organizzazioni sindacali, delle formazioni politiche della sinistra, e che anche rappresenta uno dei capisaldi di una politica di rilancio dello sviluppo anche

da un tentativo di affrontare la situazione drammatica degli incapienti (cosa che poi è stata attuata nel decreto-legge che abbiamo esaminato qualche settimana fa), nel 2008, se si determinasse una situazione nella quale a regime si registra un aumento delle entrate di tipo strutturale, la priorità nell'intervento di restituzione - su questo punto non c'è differenza tra il testo approvato dalla Commissione e la proposta del senatore Del Pennino - questa volta sarebbe da individuare nell'aumento della detrazione per le spese di produzione del reddito dei lavoratori dipendenti.

la parte marginale del lavoro autonomo, cioè le imprese che sono sotto i 30.000 euro di fatturato, riceve in questa finanziaria il più spettacolare intervento di agevolazione fiscale e di semplificazione che si sia realizzato nel corso degli ultimi decenni. È noto, signor Presidente, che alcune grandi associazioni di categoria, note per avere uffici di servizi particolarmente attrezzati, hanno calcolato che vi saranno significative eccedenze di manodopera nei loro centri servizi, determinate dal fatto che un milione di imprese grazie a questa norma non ricorreranno alle loro prestazioni. È vero che quella norma non riduce direttamente le tasse, ma nel bilancio di un'aziendina che sta sotto i 30.000 euro di fatturato, signor Presidente, colleghi, che quello che si paga si debba pagare di tasse o che si debba pagare alla società o al consulente che fa i conti per arrivare a pagare le tasse

Credo, quindi, che non si possa in alcun modo parlare di atteggiamento discriminatorio della maggioranza tra lavoratori dipendenti, che verrebbero potenzialmente premiati premiati nel 2008 se si determinerà un extragettito, e lavoratori autonomi che verrebbero penalizzati. In finanziaria già si dispone subito l'intervento a favore dei lavoratori autonomi e, nel corso del 2008, se ci sarà extragettito, ci sarà l'intervento per l'aumento della detrazione per le spese di produzione del reddito per i lavoratori dipendenti. Francamente mi sembra una soluzione equilibrata e - mi

l'emendamento 1.2 è di una rilevanza talmente enorme che supera il totale delle risorse movimentate dall'intera finanziaria. Come ha detto il collega Del Pennino, si fa riferimento all'importo che quest'Aula voterà pari a più di 425 miliardi di euro come previsione del totale delle entrate dello Stato per il 2008. Poiché questo importo è palesemente sottostimato e truccato per 14 miliardi di euro, quello che stiamo discutendo su questo emendamento e sulla destinazione di un extragettito (il tesoretto 2008), facilmente calcolabile già oggi, supera l'intera finanziaria. Qualunque cosa discuteremo da qui alla fine sarà di un importo inferiore rispetto alla destinazione di questo extragettito. È per questo che le indicazioni degli emendamenti 1.2 e 1.800 sono cruciali ai fini di una corretta restituzione di un extragettito già oggi stimabile in 13 o 14 miliardi di euro ai contribuenti che saranno chiamati a pagarlo. Per questo Alleanza Nazionale voterà a favore di entrambi gli emendamenti. Presidente, il presidente Morando ha dedicato molto tempo e molta passione

da una condizione materiale di maggiore difficoltà, quella degli incapienti. E invece, con il testo proposto dalla Commissione, si preferisce profilare il lavoro dipendente,

da parte di una maggioranza che si farebbe carico dei problemi sociali più gravi presenti nel Paese, l'aver dirottato risorse da chi sta peggio a chi sta un po' meglio.

Presidente, l'articolo 1 è di fondamentale importanza, come è di tutta evidenza, non soltanto per il significato particolare del comma 1, laddove è determinato

siano variati gli obiettivi di indebitamento e conseguentemente si proceda alla variazione dei saldi

per la tutela e la sicurezza del Paese. Sappiamo benissimo, però, che la norma è stata poi non soltanto utilizzata, ma stravolta nel suo significato nel momento in cui, in corso d'anno, sono stati variati gli obiettivi di indebitamento,

c'è ancora di più. La variazione è stata apportata in corso di discussione in Commissione e per essa il senatore Morando ha dovuto intervenire

dei lavoratori dipendenti. Il senatore Morando, cercando di convincersi, ha sostenuto che si fa questo perché all'interno dell'articolato è contenuta una serie di miglioramenti che

di grande rilevanza per il programma di politica economica della maggioranza e del Governo, la diminuzione delle tasse nei confronti dei lavoratori dipendenti. Cosa c'è di più marcatamente ideologico e classista?

un'azione pervicace e insistente con cui continua a mettere le mani nelle tasche degli italiani per prelevare quelle risorse e per darle soltanto ad una parte del Paese, i lavoratori dipendenti. Questo non possiamo accettarlo, signor Presidente. È un modo di comportarsi assolutamente classista, statalista e condizionato da quella sinistra, che vorrei definire a questo punto reazionaria, perché così opera rispetto a come il Paese vorrebbe essere governato, vale a dire con la prudenza e guardando agli obiettivi del mondo occidentale.

contraria non soltanto all'impostazione di fondo che l'UDC cercava di dare a questa finanziaria per una maggiore attenzione al problema della famiglia, soprattutto quella monoreddito,

che riproporremo anche sulle politiche sociali e fiscali di cui agli articoli 2 e 3 che andremo a discutere, dove mettiamo al centro la questione della famiglia. Con l'emendamento 1.5 avevamo proposto di destinare le maggiori entrate a sostegno del reddito familiare, votando pertanto contro l'emendamento del relatore che invece destina soltanto ai lavoratori

con il programma che avete presentato agli elettori e che avete titolato «per il bene dell'Italia». Vi siete presentati agli elettori affermando che il centro-sinistra di Prodi avrebbe unito l'Italia

sosteniamo che, se il reddito di un lavoratore autonomo e di un lavoratore dipendente è lo stesso, lo Stato li deve trattare fiscalmente allo stesso modo. Invece, voi privilegiate la vostra base elettorale, come avete fatto distribuendo i "tesoretti" a senso unico, anche nella finanziaria, per i lavoratori dipendenti. Ma c'è di più: date un'interpretazione classista dell'articolo 1 della Costituzione. A tutti voglio ricordare il dibattito che ci fu in Costituente se l'Italia dovesse essere un Repubblica fondata sui lavoratori o sul lavoro. La sinistra di Togliatti perse quella battaglia perché l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e non sui lavoratori. Ebbene, oggi questo centro-sinistra, fortemente condizionato dall'ala comunista, ripropone una storia di cinquant'anni fa pretendendo che almeno dal lato del fisco l'Italia sia fondata sui lavoratori e non sul lavoro.

su alcuni valori fondamentali dove tutte le categorie sociali si possono ritrovare perché appunto ispirate al senso dell'unità nazionale. Sarebbe stato anche un incentivo a risolvere uno dei grandi problemi del nostro tempo: mi

che ogni euro di extragettito che si fosse registrato sarebbe stato destinato alle famiglie.

intervengo per annunciare il ritiro degli emendamenti 2.3 e 2.103 e per illustrare l'emendamento 2.800.

che, in occasione di un dibattito in Aula nelle scorse sedute che riguardava l'otto per mille non hanno esitato, a sostegno delle loro posizioni, legittime, ma da me non condivise,

sostenendo che il concetto di edificio ad uso promiscuo è particolarmente dannoso per l'erario e distorsivo per la concorrenza. Bisogna quindi anche attenersi all'indicazione della Suprema corte. L'emendamento peraltro

Questo e non altro vuole sostenere il nostro emendamento. Pensiamo che sia un principio di equità e di non violazione della concorrenza. Sosteniamo che sia un modo per dare una risposta attenta, misurata, equilibrata alle sollecitazioni che ci vengono da parte della comunità.

2.5 mira ad estendere il beneficio delle esenzioni ICI a tutti i proprietari di immobili di abitazione principale, per un semplice motivo: perché qui non è in questione il livello del reddito - come impropriamente contenuto nel testo approvato dalla Commissione - ma il fatto che, sostanzialmente, l'ICI afferisce ad un bene necessario per la vita che è la casa. La casa non muta di valore con il passare del tempo per chi la utilizza, perché sostanzialmente il servizio reso è il medesimo. Questo è il motivo per il quale abbiamo proposto anche l'emendamento

deduzioni dall'imponibile e non più di detrazioni per quanto riguarda l'imposta personale dei cittadini. Cosa avvenne infatti l'anno scorso? Con l'idea di modificare il sistema fiscale, i nostri provvidi governanti passarono da un sistema

che i contribuenti si trovavano a pagare di più di quanto avrebbero pagato mantenendo il vecchio regime. Poiché siamo dell'idea che il «nuovismo» a tutti i costi, soprattutto quando è deleterio, non sia condivisibile, penso che ritornare all'antico sistema di considerare il meccanismo delle deduzioni, anziché delle detrazioni, sia più vantaggioso per i contribuenti, oltre ad essere più chiaro e, quindi, a non richiedere la necessaria consultazione di un commercialista: questa sì, senatore Morando, potrebbe essere un'innovazione non solo per le imprese, ma per tutti cittadini, nel senso della semplificazione, ed è assolutamente da sostenere rispetto all'attuale sistema che è assolutamente non condivisibile.

la nostra proposta alternativa all'impostazione della legge finanziaria. Soprattutto, si tratta di emendamenti che tengono a cuore le esigenze della famiglia

Crediamo che, al di là della specificità delle norme di ciascuno di questi emendamenti, ne sia importante il segno complessivo. Si parla tanto di agevolare la famiglia in Italia: noi proponiamo norme concrete che

è delicata. Una cosa è abolire il tributo sulla prima casa, altra cosa è decidere che per taluni è abolito e per altri no. Questo suona francamente più come un'agevolazione e invade il campo di competenza dei Comuni. Dietro questa disputa, più filosofica che concreta, se ne nasconde un'altra molto più reale.

della platea dei contribuenti al provvedimento che potrebbe portare effettivamente a degli scompensi. Ciò ha destato allarme nei Comuni stessi. Ecco perché il Gruppo di Alleanza Nazionale ha predisposto un emendamento che va in una duplice direzione: da un lato, trasforma questa abolizione parziale in un'abolizione sulla prima casa; dall'altro lato, cerca di creare un paracadute per i Comuni, introducendo la previsione che l'agevolazione che viene data sull'ICI per la prima casa

hanno determinato, tra l'altro, un tema quasi inedito in Italia, del tutto nuovo, ossia la crescita e l'accelerazione ormai travolgente dei tributi locali e della fiscalità locale, rispetto alla fiscalità nazionale. C'è il timore che anche questa norma, che è stata un po' improvvisata e dettata da esigenze di propaganda, possa continuare ad alimentare questa crescita, che determina inoltre sperequazione nel trattamento fiscale dei contribuenti da città a città, in maniera sempre più evidente. sono sotto gli occhi di tutti. In questo momento, mentre stiamo votando, abbiamo aree metropolitane importanti, come Roma, che hanno un livello di tassazione locale doppio rispetto a quello di altre aree metropolitane simili, omogenee e con una platea di contribuenti del tutto comparabile, come può essere l'area di Milano. C'è il timore che questa crescita, alla quale peraltro non corrisponde una migliore offerta di servizi, nel senso che la variabile risulta indipendente dalla qualità dei servizi, possa, attraverso la norma così come proposta, essere ulteriormente incrementata. Questo è il senso dell'emendamento, che attraverso queste due modifiche tenta di rendere più equo lo sgravio e più sicuro l'effetto dello stesso dal punto di vista dell'autonomia dei Comuni e degli enti locali.

una contestazione volta in direzione di uno dei contraenti di questo patto è altrettanto rivolta ad una maggioranza e ad un Governo che per la famiglia e per i giovani, nonostante i proclami, non hanno fatto nulla. Per tale motivo questi due emendamenti, in particolare il 2.9, anche se toccano in modo marginale la questione, cercano di dare risposta alle esigenze che le famiglie rivolgono al mondo della politica. Voglio ricordare ancora una volta che presso la Commissione finanze del Senato giacciono disattesi i disegni di legge sul quoziente

2.9 propone di differenziare la detrazione massima ICI a seconda che il soggetto passivo sia un singolo o un nucleo familiare. È evidente che esistono situazioni

per le spese sostenute per l'affitto, l'energia elettrica e il riscaldamento. Credo che uno dei maggiori problemi delle famiglie riguardi proprio gli enormi costi che esse devono sostenere in questi tre campi

signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo UDC, con prima firma del capogruppo D'Onofrio, ha presentato diversi emendamenti sull'articolo 2.

che, insieme ad altri temi come quello dei giovani, della casa, della sicurezza, delle infrastrutture e della impresa che crea lavoro e quindi rende una famiglia dignitosa socialmente e civilmente sono stati i temi sui quali tutto il centrodestra si è ritrovato per poter presentare emendamenti con firma congiunta dei Gruppi dell'opposizione. la famiglia su questi temi figura al primo posto perché riteniamo che riassorba l'universo mondo anche degli altri temi.

non riguardano direttamente la famiglia ma situazioni marginali che possono essere ricondotte alla famiglia. Riteniamo che la maggioranza abbia voluto

aumentato le detrazioni dall'ICI sulla prima casa e, quindi, di aver dato un contributo, un sollievo ai problemi della famiglia: che per il centro-sinistra, durante il Governo del centro-destra non arrivava alla quarta settimana del mese, oggi, se dovessi stare alla stessa retorica, alla stessa demagogia della sinistra, direi che non arriva nemmeno alla terza settimana! Questo Questo emerge soprattutto dalle denunce provenienti dallo stesso mondo sindacale che fiancheggia il centrosinistra, che per non rovesciare il Governo Prodi non ha organizzato le grandi manifestazioni romane dei cinque anni precedenti, ma che comunque ha dato il segno dell'insofferenza e del disagio che i ceti sociali più deboli denunciano. Ebbene, avete dato una risposta con l'articolo 2 della finanziaria 2007 rimodulando la curva della distribuzione dei redditi attraverso un'operazione fiscale, che sostituiva le deduzioni del centro-destra con le detrazioni del centro-sinistra per redditi inferiori ai 25.000 euro. Dobbiamo constatare che, all'indomani dell'approvazione dei bilanci degli enti locali, soprattutto dei Comuni e delle Regioni che con le addizionali hanno compensato e quindi inficiato i benefici per i redditi fino a 25.000 euro,

Non solo, accanto al maggiore carico fiscale sulla famiglia, soprattutto, ripeto, quella con figli a carico e monoreddito, ci siamo ritrovati un modesto aumento degli assegni familiari, sui quali però hanno pesato gli aumenti delle tariffe domestiche (luce, acqua, gas e telefono), oltre alle tariffe

Scusi, senatore Ciccanti. Pregherei i colleghi di abbassare il volume della voce, altrimenti il senatore Ciccanti non può sviluppare il suo importante intervento,

le norme Visco, molto più pregnanti e sostanziose di quei decreti e che creavano un maggiore carico fiscale e maggiori adempimenti fiscali per gli italiani. Ecco, noi oggi in questa finanziaria siamo necessitati ed obbligati, sentiamo su di noi un peso non solo politico ma anche morale, a riproporre la centralità del tema e della famiglia; lo abbiamo fatto già nella passata legislatura con i Governi Berlusconi ed a maggior ragione lo rifacciamo con voi. è già stato detto da chi mi ha preceduto: non c'è una norma che riguardi direttamente la famiglia dal punto di vista fiscale.

perché è particolarmente odiosa per coloro che stanno pagando un mutuo per la prima casa e perché la riduzione di questa tassa determinerebbe una maggiore disponibilità di reddito per l'86 per cento degli italiani, che potrebbe essere destinata ai consumi interni, che si sa essere la voce principale per il rilancio dell'economia.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione dicendo che avevamo proposto anche per l'emersione dal nero

senatore Pollastri, vi pregherei di accomodarvi, perché il brusìo è insopportabile, i colleghi oratori hanno difficoltà ad esprimersi. Pregherei i colleghi di prendere posto. Chi deve parlare può accomodarsi fuori dall'emiciclo.

italiane, quelle che, in stragrande maggioranza, hanno acceso un mutuo a tasso variabile. Di fronte a questo problema il Governo e la maggioranza che lo sostiene propongono una soluzione assolutamente inadeguata;

quando fu portato quel limite a 7 milioni delle vecchie lire; ebbene, quei 7 milioni sono rimasti 3.500 euro in quarant'anni di vita repubblicana. Voi, con un'operazione che è solo uno *spot* senza alcuna sostanza, aumentate quel limite da 3.500 euro a 4.000 euro, ma su di esso verrà applicata l'aliquota del 19 per cento; il risultato di quest'operazione sarà che voi darete ad una famiglia italiana che ha acceso un mutuo a tasso variabile una detrazione fiscale netta di 70 euro annui, corrispondenti a 5,6 euro mensili. Questo è il risultato della vostra operazione! Voi non comprendete i problemi che stanno vivendo le famiglie italiane in conseguenza del rialzo dei tassi d'interesse che si sono scaricati sulle rate dei mutui per importi che sono dell'ordine di oltre 1.000, 1.200 euro annui, e voi rispondete con 70 euro di detrazione fiscale.

mi rivolgo al senatore D'Amico, che pure si è fatto carico di questo problema in Commissione finanze, mi rivolgo ai tanti senatori che sono nell'Ulivo, senatore Bobba, alla senatrice Binetti, che hanno condiviso la necessità di un intervento più robusto per le famiglie. Non potete pensare di aver risolto il problema con un intervento così irrisorio rispetto alla gravità di una situazione che richiede ben altra assunzione di responsabilità. Vi chiediamo di non prendere in giro le famiglie italiane; vi chiediamo un atto di responsabilità!

attraverso il superamento del cuneo fiscale, un'imposta sulle rendite finanziarie e una riduzione di spese militari, al fine di costruire un vero risarcimento sociale. Mi riservo brevi dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti e dichiaro fin d'ora il mio sostegno all'emendamento 2.800 del senatore Montalbano, analogo al mio

manca la percentuale di aumento dell'ICI sulle case sfitte, che dovrebbe essere fissata in modo tale da rendere l'emendamento coperto. Ovviamente i 400 milioni

con mio grande stupore, salvo poi ritrovarlo identico e preciso in un emendamento del relatore all'articolo 5.

Inoltre, voglio aggiungere che questo Governo si era assolutamente dimenticato di inserire la detassazione del lavoro frontaliero nella prima stesura.

Sarà un caso che questo Governo abbia dimenticato, nella prima stesura, una detassazione parziale del lavoro frontaliero? Questa fu un'invenzione nel 1999 dell'allora presidente del Consiglio Amato, che, raschiando il fondo del barile, si mise a tassare persino i redditi da lavoro frontaliero. Guarda caso, l'onorevole senatore Amato oggi fa parte di questo Governo ed è Ministro dell'interno, potenza delle coincidenze.

Credo che questa sia davvero una situazione kafkiana, che punisce - torno a ripeterlo - gente che va a lavorare all'estero tutte le mattine perché non trova lavoro a casa propria e che, soprattutto, in qualche maniera porta valuta a casa nostra. Nonostante il relatore abbia accolto *a posteriori* il mio emendamento, prima respingendolo, poi facendolo proprio, pur senza il mio nome, ribadisco che lo ringrazio. Gli chiedo però di valutare con attenzione

signor Presidente: mi rivolgo non all'Aula, ma ai pochissimi che hanno ancora voglia di ascoltare; poi, però, farò anche riferimenti personali. Il primo emendamento che vorrei illustrare è il 2.72. Partiamo da una riflessione: il Governo sta varando

tutta la sicurezza che viene dalla domanda sociale. Cosa fanno i cittadini, se lo Stato non sa offrire la sicurezza adeguata? Si «attrezzano», si autoproteggono: sempre di più, sistemi di protezione per le abitazioni (pensiamo a porte blindate, a finestre di sicurezza ma anche a sistemi di allarme) non sono un vezzo, ma stanno diventando quasi una necessità. Necessità contrapposta alla carenza di capacità, da parte delle strutture pubbliche, di tranquillizzare e rendere la vita più serena. Riteniamo corretto che lo Stato consenta una detrazione su tutti i materiali di edilizia comunque destinati a garantire la sicurezza degli edifici paragonata a quanto sta facendo per chi fa interventi che risparmio energetico: chiunque faccia interventi per attutire l'impatto dei consumi energetici riesce infatti ad ottenere una detrazione del 55

stortura del sistema? Nel momento in cui percepisce questo trattamento di fine rapporto anche per redditi medi‑medio bassi,

Il nostro emendamento prevede, quanto meno, una fase di mediazione: una tassa fissa che non superi il 18 Pensiamo, colleghi (mi rivolgo soprattutto ai più sensibili della sinistra), che le rendite finanziarie sono tassate al 12,5 per cento: non è possibile che un reddito da lavoro, percepito nel momento "x" ma accumulato ma accumulato nell'arco di una vita, venga tassato in modo più gravoso di una rendita finanziaria. Quel 18 per cento potrebbe essere un segnale per far capire che non si va sempre a spremere dove forse ci sarebbe da redistribuire. Per i colleghi della sinistra che l'hanno capito, ringrazio.

riconosceva la ruralità di tutti i fabbricati delle cooperative e dei consorzi adibiti alla trasformazione di prodotti agricoli.

approvare questo emendamento,

sostenere l'emendamento 2.0.31 - che per la verità ricalca le linee di un disegno di legge che ho già presentato, ma che verrà in discussione in tempi molto più avanzati

ma capisco che non a tutti piaccia andare a disturbare la Banca d'Italia, che invece, alla muta e alla sorda, fa finta che questi soldi siano suoi.

e per i premi aziendali, vale a dire quel lavoro che nelle nostre aziende viene svolto spesso fuori

condizioni. Crediamo che con questo emendamento si possa sostenere e aiutare il miglioramento della retribuzione media dei lavoratori,

del rinnovo del contratto, la FIAT ha iniziato una nuova politica delle retribuzioni. E allora, ancora una volta, è forse la politica, sono forse le istituzioni, ad arrivare tardi rispetto ad un processo regolato fortemente dal mercato, nel quale dobbiamo entrare il meno possibile dal punto di vista del peso aggiuntivo. Questo è il motivo per cui riteniamo fondamentale riuscire ad affrontare e poi colmare - ci auguriamo - il divario che sta crescendo tra noi e gli altri Paesi europei in tema di salari. Pensiamo che, ricollegandosi alla produttività

disposto a scommettere sulle proprie capacità, sul proprio talento e sulle proprie aziende al fine di aumentare la produttività. Cito un ultimo dato, perché si possa comprendere ancora meglio questo fattore

sui grandi valori della formazione, della flessibilità e del lavoro, ha potuto sviluppare *performance* straordinarie. Tentiamo Tentiamo dunque di fare la nostra parte, cominciando a detassare in modo sensibile la scommessa che i lavoratori e gli imprenditori del Paese devono poter fare sulla produttività.

in modo tale da poter poi esprimere i pareri senza motivarli ulteriormente. La Commissione ha ritenuto, in accoglimento di un emendamento

e castelli, in tal modo eliminando l'intralcio burocratico e gli adempimenti connessi all'onere della dimostrazione della possidenza di un reddito inferiore ai 50.000 euro. Inoltre, si è provveduto a precisare le modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni. Tutti gli altri emendamenti vanno in senso opposto opposto alla decisione assunta dal Governo con il testo originario e a quella della Commissione, poiché propongono soluzioni alternative che determinerebbero scelte diverse e più diverse e più problematiche, ad esempio in ordine alla possibilità di trasformare questa detrazione in detrazione IRPEF.

tratta il tema noto dell'ICI sugli immobili di proprietà delle confessioni religiose, compresa quella cattolica, e di altri enti non lucrativi,

versa sullo stesso tema, anche se relativamente ad una nicchia di immobili, ossia i padiglioni e le aree fieristiche, chiedendone la riclassificazione. Non se ne comprende la ragione, quindi esprimo parere contrario.

2.500 propone la detrazione dell'ICI dall'IRPEF: nuovamente, non vi sarebbero argomenti di principio contrari, ma è inaccettabile la copertura, che si ricava con l'aumento dell'imposta di bollo. Torno a sottolineare che con questa finanziaria non aumentiamo neanche un euro di imposte, tariffe o tasse, il che, appunto,

dell'ICI sulle case sfitte e su altri immobili indicati: mi riferisco alla precisazione fatta dianzi del 10 per mille sostitutivo, appunto, del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI per la prima casa. A mio modo di vedere, i problemi sono tanti per un norma di questo tipo: vi sarebbe una sperequazione notevolissima a sfavore delle tipologie di immobili indicate ma, soprattutto, vi è un problema di congruità della copertura. È stato stimato che per l'abolizione dell'ICI per la prima casa occorrono almeno 2,4 miliardi di euro. Questo emendamento reca una copertura di soli 400 milioni

di esprimere una propensione favorevole a una norma di questo tipo, che costituirebbe una formidabile leva per l'emersione del nero e del sommerso relativamente ai redditi da locazione. La copertura di una norma di questo tipo è tuttavia molto complessa. Si è stimato che per adottare una misura di tale genere occorrerebbero almeno 1,5 miliardi. Fermo restando l'impegno, inviterei i proponenti, se lo ritengono, a predisporre un ordine del giorno. Credo che né la maggioranza né il Governo avrebbero difficoltà a considerare un impegno di questo tipo anche nel contesto della riforma delle rendite finanziarie (vi è infatti una certa similitudine tra i

caso, inviterei i senatori D'Onofrio, Ciccanti e gli altri colleghi del Gruppo dell'UDC, se lo ritengono, di presentare un ordine del giorno. Ci sono infatti problemi di copertura e di valutazione della congruità di una norma di questo tipo con il sistema delle detrazioni sugli affitti introdotto dall'articolo 2. Esprimo

cento dell'importo vigente. Stante la necessità, anche qui, di provvedere a una copertura significativa, riteniamo che il passo importante che è stato fatto in Commissione

l'estensione delle tipologie di spesa familiari deducibili dal reddito. Naturalmente questo tema incide sul sistema delle deduzioni e delle detrazioni necessita di una copertura finanziaria ragguardevole, tant'è che si provvede a coprirlo riducendo quell'anticipazione finanziaria a favore delle Regioni in condizioni di dissesto sanitario,

perizia sul valore dei terreni e un'imposta sostitutiva nella cessione di aree e immobili indicati nell'emendamento. Per

un parere favorevole. L'emendamento 2.72 tende ad accrescere la detrazione per la ristrutturazione degli immobili dal 36 al 55 per cento relativamente a talune spese, in particolare quelle per la sicurezza degli edifici.

emendamenti 2.0.500, che tende a reintrodurre la scala mobile per il dipendenti pubblici, pubblici, e 2.0.4, che affronta il tema delle pensioni minime e massime con coperture relative alla tassazione delle transazioni valutarie che allo stato sarebbe molto complesso valutare

Invito a ritirare l'emendamento 2.0.10 perché il tema è ampiamente affrontato nel modo che potrà verificare con la riformulazione dell'articolo 91 (emendamento Villone ed altri);

in Commissione: il senatore Vegas e gli altri senatori propongono di rafforzare il pacchetto casa, già consistente e corposo, mediante una misura innovativa, ovvero destinare le risorse Sviluppo Italia ad un fondo rotativo, finalizzato alla costruzione di case. Il problema è verificare l'esistenza e la congruità delle risorse, tema che potremo affrontare nel futuro. Inviterei i colleghi a valutare eventualmente la presentazione di un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

far notare all'Aula e a codesta Presidenza che anche se certamente, a termini di Regolamento, non si può obbligare il Governo a rendere un parere un po' più esteso rispetto ad una succinta dichiarazione di conformità, avrebbe fatto onore, non soltanto all'Aula ma anche al relatore, un parere del Governo un po' meno

Chiedo però formalmente al Ministro dell'economia di far avere all'Aula una lettera firmata dal sottosegretario Sartor per garantire le coperture che il senatore Legnini ha messo in dubbio. Senatore Baldassarri, questa sua sollecitazione l'abbiamo ascoltata ripetutamente e lei tenacemente la ripropone. La Presidenza non può far altro che prendere atto di questa sua sollecitazione; il Governo ha facoltà di parlare o meno, come lei ben sa.

che ci si è venuti a dire in modo apodittico che ci sarebbe la copertura. È però tradizione di questo e dell'altro ramo del Parlamento che quando la finanziaria, passato l'esame delle Commissioni, arriva in Aula essa sia correlata da una relazione tecnica

questi due colleghi, autorevolissimi e competenti, pongono tale questione. Ho già avuto modo di dir loro in Commissione che dopo che hanno votato un emendamento con 2 miliardi di copertura sui fondi perenti farebbero meglio a stare zitti.

intervenuti, ma le ragioni addotte dai colleghi Vegas e Baldassarri non sono questioni di lana caprina, perché attengono al regolamento di contabilità dello Stato ed anche ad un imbarazzo evidente della maggioranza,

che apprezziamo per le modalità con cui si rapporta in Commissione, ma non per questa mania di fare le pulci all'opposizione, di dare patenti di moralità oppure di invitarci al silenzio: ricordo che questo è un Parlamento e che l'opposizione ha tutti i diritti di votare quello che le sembra opportuno, senza chiedere il permesso preventivo al collega Boccia o a chicchessia. *(Applausi

una famiglia in cui il marito ha a carico la moglie ottiene una detrazione familiare di 100 euro, la stessa detrazione viene presa da un *single*. Con l'emendamento 2.9, cerchiamo di di evidenziare che le famiglie con moglie a carico o con più figli hanno diritto a più detrazioni. Faccio presente che oggi il maggior rischio di povertà non è tanto dato dall'esclusione sociale, ma dal numero di figli:

Presidente, ritengo che le argomentazioni addotte

è che non si può nascondere, senatore Legnini, la testa sotto la sabbia anche quando c'è un'ingiunzione da parte comunitaria rispetto all'esenzione dell'ICI sui locali commerciali delle ONLUS e delle confessioni religiose. La Comunità ha dato 30 giorni di tempo al Governo italiano per rispondere su questa materia. Il Parlamento italiano è nelle condizioni oggi di esprimere una sua valutazione, un suo intendimento, una sua posizione su tale questione. Tuttavia, mi pare che serpeggi nella nostra Aula una sorta di invito garbato e suadente ad una disciplina di maggioranza, rispetto anche a temi di questa natura. Signor Presidente, mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che riterrei comprensibile un invito alla disciplina di maggioranza laddove fosse indirizzato all'integrità della manovra finanziaria,

mi chiedo - e chiedo ai tanti colleghi che legittimamente sono contrari e ai tanti colleghi che legittimamente possono essere favorevoli su questo emendamento - se non sia il caso

Non comprendiamo, quindi, la chiamata alle armi e a far quadrato su questo emendamento. Vi è una prima questione che riguarda il pronunciamento della Comunità.

come giustamente sostiene la Comunità, l'applicazione di questa norma. Ebbene, nonostante la Corte di cassazione dica ciò, noi invochiamo il principio della disciplina di maggioranza; lo invochiamo in una strana continuità, onorevole Presidente,

Ecco qual è il punto su cui vogliamo richiamare l'attenzione; vogliamo anche invitare i colleghi che hanno sempre fatto della laicità una bandiera della loro appartenenza, della testimonianza della propria battaglia politica e della propria identità politica e culturale

elettronico. Chiediamo a quanti colleghi hanno coerentemente ribadito e sottolineato il consenso attorno a questi temi di manifestarlo nel voto.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la questione posta dal collega Montalbano con questo emendamento è parte di una discussione molto importante,

Desideriamo che in quest'Aula si faccia chiarezza in modo preciso sull'intendimento del Parlamento nei confronti di un emendamento che è figlio della peggiore cultura laicista e di chi non conosce la storia del nostro Paese. Leggo l'emendamento, perché non ha nulla a che vedere con il voto dei cattolici, ma con quello degli italiani, sensibili al fatto che l'assistenza non è riserva di questa o quella parte politica, ma un bene comune del Paese. Vogliamo che in questo Parlamento la maggioranza, larga, si esprima al di là dell'appartenenza cattolica o meno dei singoli senatori, perché non è in gioco una questione di fede, ma di pura laicità dello Stato. Leggo l'emendamento, perché probabilmente non è stato capito fino in fondo che con esso non è in gioco la laicità dello Stato, ma la pretesa di sottrarre anche le opere destinate alla beneficenza espressamente non a fini di lucro

penso che i colleghi lo sappiano - che l'Unione Europea abbia mai contestato al Governo italiano una norma del genere. Ritengo un fatto di grande significato il decreto del Governo Berlusconi e che Bersani lo abbia confermato. È la prova che su questa questione non ci si divide per schieramenti politici, né tra laici e cattolici, ma tra tutti quelli - che mi auguro siano la maggioranza, sempre più larga - che sono interessati a veder salvaguardate queste istituzioni,

non è vero che l'Unione Europea abbia mai contestato alcunché; ha chiesto chiarimenti al Governo italiano, cosa totalmente diversa dalla procedura d'infrazione. Non è vero che la Cassazione abbia dichiarato questa norma illegittima, ha invitato a prestare attenzione ai problemi della concorrenza: sono due cose radicalmente diverse. I colleghi sono capaci di intendere e di volere e il voto elettronico dimostrerà - come sono convinto - che essi sono contrari all'emendamento, per ciò che esso dice. Lo leggo, nell'eventualità che non sia stato compreso fino in fondo.

«l'esercizio di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro». Non si agevolazioni ICI il fine di lucro, ma dell'ipotesi, che il laicismo deteriore per molti anni ha imposto a questo Parlamento, di sottoporre a regole vessatorie le nostre istituzioni caritatevoli e di buona volontà.

Signor Presidente, svolgo questa breve dichiarazione di voto a nome dei Gruppi di Rifondazione Comunista, Insieme per l'Unione e Sinistra Democratica. Noi condividiamo il contenuto dell'emendamento 2.800 e lo condividiamo ancora più fortemente dopo aver udito l'intervento del collega D'Onofrio. Riteniamo che, come ha già dichiarato il collega Montalbano, si tratti di un atto quasi dovuto rispetto alla normativa europea, che peraltro ci chiamerà presto di nuovo a misurarci su questo terreno. Svolgiamo anche una considerazione sul contenuto di questo emendamento e rispetto alla questione di fondo che esso richiama, che è la

contro ogni privilegio concesso non alla fede religiosa, non alle coscienze religiose, ma al potere istituzionale e alla libertà di commercio di una grande, pur rispettabilissima istituzione, come la Chiesa cattolica. Tutte queste ragioni, che sarebbe necessario, certo, discutere molto più a fondo perché hanno una lunga e complessa storia alle spalle, ci porterebbero naturalmente a votare a favore di questo emendamento. Tuttavia, noi non faremo questa scelta per ragioni di natura strettamente politica. Noi abbiamo lavorato, in questo ramo del Parlamento, abbiamo raggiunto un equilibrio sul testo di questa manovra finanziaria che è costato lunghe discussioni e che ha coinvolto tutte le forze della coalizione, producendo un risultato importante, unitario e soddisfacente. Per tutte queste ragioni esprimiamo qui una scelta di astensione di cui, signor Presidente, vorrei fossi chiaro il valore politico. Anche se sappiamo che tecnicamente il voto ha valore diverso, politicamente per noi questo è un voto che ci costa molte difficoltà, è un voto sofferto, perché la nostra propensione ci spingerebbe ad esprimere un voto favorevole.

Tuttavia, il senso di responsabilità in questo momento ci fa esprimere questa - ripeto - sofferta scelta. Mi auguro che un analogo senso di responsabilità, nella lunga strada di votazioni che ci aspetta, sia diffuso in tutte le componenti della coalizione.

che erano alla base dell'accorato appello del senatore Montalbano (che condivido pienamente), voterò a favore di questo emendamento.

non risponderanno positivamente all'invito non garbato ma provocatorio del contenuto dell'emendamento. Lo dico per ragioni di merito e di principio. Il merito sta nelle parole pronunciate poc'anzi dal presidente D'Onofrio: anch'io sono rimasto basito dalla lettura testuale dell'emendamento scritto e presentato dal senatore Montalbano. Pensavo di aver sbagliato io nella lettura, pensavo ci fosse un errore di stampa, ma il fatto che ci sia un'autorevole opinione, ben più importante della mia, come quella del presidente D'Onofrio, mi conforta nella lettura esatta, nell'interpretazione autentica - non da parte di Bersani ma da parte di tutti noi - delle scempiaggini che sono scritte in questo emendamento. Quando si afferma che «l'esercizio di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta comporta la decadenza dal beneficio», vuol dire che si ha nel mirino un'istituzione morale di questo Paese e credo non sia accettabile oggi in Italia avere ancora questo tipo di argomenti in testa.

ci consentirà di spiegare al Paese che non è vero che ci debba essere rassegnazione verso la pretesa di cancellare ogni traccia di presenza delle attività sociali della Chiesa nel nostro Paese.

Collega Montalbano, voi vi ponete il problema di quello che fa la Chiesa e non vi rendete conto che la gente si pone il problema di quello che vengono a fare i profeti di altre religioni nel nostro Paese.

Al Parlamento, al Senato, alla Casa delle Libertà, alle persone che non vogliono cedere chiedo modestamente di dare un segnale vero di fierezza di un'identità contro un emendamento che invece è un pessimo segnale verso la Chiesa e verso la comunità nazionale. Per fortuna, ho la speranza che il Parlamento, senatrice Gagliardi, proprio nella sua sovranità, respinga questa proposta sconcia.

i Popolari-Udeur voteranno contro l'emendamento 2.800 in materia di esenzione fiscale ICI. Prendiamo atto dell'atteggiamento della sinistra su questo punto e di conseguenza ci sentiamo liberi di comportarci in maniera analoga nella prosieguo dell'esame della legge finanziaria. *(Applausi Signor Presidente, sarò molto breve perché il collega D'Onofrio ha già spiegato in profondità i motivi per i quali

ha il dovere politico di non approfittare della distrazione dell'Assemblea nel farlo, ma di motivarne le ragioni. La mia ragione non è neanche tanto ideologica, come ho sentito affermare in altri interventi,

di cui si occupa l'emendamento in discussione, chiama in causa attività ricettive, sportive, ricreative e così via che possono essere svolte, pur senza fini di lucro, anche da istituzioni non religiose.

per la concorrenza. Non mi risulta che il Commissario europeo per la concorrenza abbia competenze ed interessi di carattere ideologico; credo si occupi di aiuti alle imprese commerciali e della loro legittimità, come - appunto - nel caso in questione.

molto delicati e comportino per tutti noi un'assunzione di responsabilità, intanto nel rispetto di tutte le sensibilità e di tutte le visioni.

Mi sembra giunga un messaggio che sottolinea divisioni. Ma perché? A quale fine? Qual è il risultato operativo che si porta a casa con l'approvazione di questo emendamento, con il sottolineare divisioni?

di estrema cortesia verso le differenti sensibilità che sono rappresentate in quest'Aula e in questa maggioranza. Non v'è chi non veda che la proposta che deriva da questo emendamento è francamente schizofrenica. Ora, indipendentemente dalla formulazione letterale e tecnica del testo, e non chiamerei a giustificazione né l'Unione Europea né la Corte di cassazione

italiane, dove gli oratori funzionano da aggregazione per togliere dalla droga ragazzi e giovani di paesi, città e metropoli. Proprio perché non siamo più in questa lettura, cioè in una lettura ideologizzata delle posizioni, vediamo lo scopo finale. Lo scopo finale di questo emendamento crea solo divisioni.

proposta, nella vostraidea, non ci sia questo, ma lei, senatore Montalbano, mi insegna che questo è il messaggio che ne deriva e questa è la polemica politica che poi ne scaturisce. Ne sono esempio

non siamo in una visione di rapporto estremamente superato, un po' da 1870, di Stato contro Chiesa. Siamo in una funzione e in una visione storica nuove, diverse. Siamo nel 2007, senatore Montalbano. Siamo in una realtà quale probabilmente la lucidità di questo Parlamento, la lucidità di quest'Aula, ha portato il senatore Legnini a fare questa proposta. Sarebbe un grande segno di saggezza, mantenendo le opinioni che i sottoscrittori hanno, accettare questo invito al ritiro, lasciando aperto l'argomento.

il problema delle esenzioni ICI per gli istituti religiosi e le costruzioni annesse e non principali è stato già affrontato nella passata legislatura e risolto, anche in considerazione del fatto (quando fu proposta la norma non fu coperta) che la difficile interpretazione della disposizioni già vigenti nel 2004 aveva

Sottolineo questa sua capacità politica di presentare emendamenti innocui e ritirare magari quelli pericolosi. Al di là di questo, rivendico il il fatto che l'esenzione ICI venne introdotta dal nostro Governo. Lo riteniamo un fatto di cui menare vanto, perché badate che qui ci sono colleghi molto più giovani di me, ma io sono uno di quei ragazzi cresciuti in un'Italia che forse era anche migliore di questa, quando c'era la Topolino, non c'erano palestre, né campi sportivi, e giocavamo a pallone sulla ghiaia degli oratori. Non bevevamo la Coca-Cola, ma la spuma, e mangiavamo la liquirizia tagliata a stringhe che compravamo nel baretto dell'oratorio.

di *revival* in quest'Aula: sembra di essere tornati ai tempi ottocenteschi con questa divisione fra clericali e anticlericali, perché è evidente che c'è una connotazione ideologica in tutto ciò. voterò contro questo emendamento, ma riconosco anche che è un emendamento che riguarda più le coscienze che la politica. Quindi, il Gruppo della Lega voterà secondo coscienza, ciascun senatore regolandosi come crede.

assolutamente legittime, fosse rivolto alla parte dell'emendamento che recita: «e non sia rivolta a fini di lucro».

l'espressione «e non sia rivolta a fini di lucro» oppure se la cancella. Non può subordinare questa seconda eventualità alla possibilità di un cambiamento di opinione politica, parlamentare e di voto da parte dei colleghi. Lei mi deve dire che cosa

Questo vuol dire forse che l'emendamento originario s'intende decaduto e quindi riformulato? Se si intende che egli abbia rinunciato, lo faccio mio per metterlo ai voti e farlo bocciare.

contro la riformulazione, ma non vogliamo lasciar passare il principio che attraverso un trucco si possa tentare di fare rientrare dalla finestra ciò che è stato mandato via dalla porta. Ritengo che ne abbiamo diritto, Presidente, e lo dico anche per una questione di equilibrio che riguarda lei stesso, che è tra i firmatari dell'emendamento. Evitiamo interpretazioni forzate rispetto a un emendamento che è chiarissimo. Se lo si vuole votare per parti, lo si chieda all'Aula. L'Aula si pronuncerà se è d'accordo alla votazione per parti separate, ma non credo che ciò sia più nella sola disponibilità

prendete di nuovo. La vostra schizofrenia è il motivo per cui avete perso il consenso del Paese. La vostra schizofrenia fiscale è il motivo per cui proponiamo di votare questo emendamento ed insistiamo affinché con la sua approvazione si realizzi ciò che cerchiamo di fare, una vera rivoluzione nel Paese. Senatore Giannini, ci dispiace, ma è oggi l'anniversario della Rivoluzione di ottobre.

Con esso si determina una moratoria rispetto a quanto sta accadendo negli accatastamenti. Migliaia di lettere sono giunte ai cittadini contribuenti di Napoli

dalle migliaia di lettere che stanno giungendo ai contribuenti. È assolutamente necessaria una moratoria per fare il punto della situazione.

favorevole perché, a nostro avviso, l'emendamento 2.23 del senatore Eufemi entra nel vivo di una delle questioni economiche e finanziarie che destano molto allarme negli ultimi tempi, quella dei mutui. Penso che il tempo manchi in questa sede, in questa occasione per richiamare alla nostra attenzione la grande partita della crisi dei *subprime* che ha scosso i mercati finanziari internazionali. Però, va da sé che che dobbiamo prendere atto del fatto che il peso dei mutui sta gravando ogni oltre misura ed oltre un limite accettabile sulle famiglie italiane, soprattutto quelle che avevano sottoscritto mutui a tasso variabile e che si ritrovano oggi la spiacevole sorpresa di vedersi pretendere dalle banche rate sempre più esose e non hanno spesso la possibilità di diluire ulteriormente nel tempo il peso di queste rate. Ecco allora che l'emendamento punterebbe intanto a rivedere quell'aliquota

godere almeno di un beneficio fiscale, così come prendiamo atto del fatto che per questo Governo la somma di

il limite che segna come un argine insormontabile tale questione.

messo in evidenza un tema che il relatore prima stentava a comprendere. Quando il relatore si è chiesto la ragione di un emendamento che potesse ulteriormente agevolare il sistema fieristico italiano dal punto di vista dell'ICI, quello che suggerisco al relatore è di chiedere a qualche fiera italiana,

di vista, aiuterebbe loro a sostenere quel processo di *marketing* tanto utile alle nostre imprese che il sistema fieristico garantisce.

essendo estranea per materia l'emendamento al 2.23.

Presidente, ringrazio la senatrice Bonfrisco. Questa norma è assolutamente interpretativa rispetto agli orientamenti dell'Agenzia del territorio che tende ad attrarre gli immobili adibiti a padiglioni fieristici nella categoria catastale D8. D8. Sappiamo che questo non è un problema di centro, di destra o di sinistra. Esso riguarda Verona come Palermo, Milano come Bari, Roma come Milano. E' un problema di dare il significato giusto alle fiere che

funzione economica. Quindi, è soltanto una norma interpretativa rispetto agli orientamenti del Ministero delle finanze. Mi auguro che l'Aula superi steccati tra maggioranza e opposizione e trovi il modo di risolvere un problema che riguarda tutto il *made* *in* *Italy* e gli operatori delle piccole e medie imprese.

la relazione tecnica sull'intera manovra della legge finanziaria. Si tratta di una copia che riporta la data del 6 novembre, giunta alla Commissione mezz'ora fa, in data 7 novembre. La lettera di trasmissione è a firma del capo di Gabinetto del Ministero Paolo De Ioanna e le tabelle e la relazione sono firmate dalla Ragioneria generale dello Stato. Stato. Ho il dovere di informare l'Aula che in queste tabelle, nell'ultima parte, è scritto con precisione: «Effetti da recuperare in sede di coordinamento o modifiche con emendamenti tecnici delle seguenti norme». Guarda caso, si tratta della norma sui *ticket.* Quindi, quest'Aula, prima di votare, deve

**Il Senato non approva.**

si verificano questi comportamenti da parte di banchieri militanti nel Partito democratico della sinistra e, all'interno di quello schieramento, nessuno avverta l'esigenza morale di prendere le distanze da questo autentico scandalo? Si tratta di vera e propria usura. Non è possibile che il cliente della banca che risiede in Olanda paghi all'Unicredit un interesse inferiore del 40 rispetto a quello pagato dal cliente italiano. E poi venite in televisione a dire che non si arriva alla fine del mese. Dovete ringraziare Iddio che l'informazione dei

e la televisione siano espressione di questi poteri; che la stessa Gabanelli su RAITRE sia espressione di questi poteri, perché mente su queste cose, omette questi autentici scandali del sistema bancario italiano.

Presidente, riallacciandomi agli interventi precedenti vorrei manifestare il mio stupore riguardo al comportamento non di un Governo, ma di una maggioranza che sul tema dei mutui sta dimostrando un totale appiattimento sulle politiche bancarie dei grandi gruppi d'Italia; politiche che si rifanno ad una logica sostanzialmente coerente rispetto a quella adottata dal Governo sostenuto da questa maggioranza

hanno goduto di estremi vantaggi dal punto di vista politico e mediatico. Quindi, non ci stupisce che il Governo lo sia, ma ci stupisce la sensibilità di una maggioranza che, invece, dovrebbe apprezzare quanto fatto dall'opposizione, in particolare con questo emendamento del senatore Eufemi, e dalle politiche che Alleanza Nazionale svolge sui mutui in ogni parte d'Italia. Dove sono gli animi, vicini ai lavoratori, di coloro i quali dicono di difenderli? Si ha un bel da fare oggi a propagandare posizioni contro la Chiesa in maniera vergognosa

perché i mutui intervengono in maniera pesante. Cosa vogliamo fare? Vogliamo mettere in ginocchio una categoria, quella dei lavoratori italiani e dei piccoli impiegati, i quali non arrivano a pagarsi la rata di mutuo e vedranno questa loro condizione esasperata fino a perdere quel bene al quale agognano da una vita intera?

che - come diceva bene un rappresentante della Lega - ci ricorda i nostri tempi giovanili, nei quali quasi tutti abbiamo calcato le spiagge o i campi dei salesiani o di altri ordini religiosi. Questa sinistra, così feroce contro questo tipo di istituzione, che tanto bene fa alla società,

ma sicuramente i piccoli cittadini, che da questa grande finanza sono fortemente lontani, per fortuna loro.

subito. Mi fa piacere che siano presenti il Ministro della giustizia ed un rappresentante del Ministro dell'economia. Abbiamo formulato un emendamento, spiegando che l'aumento dei mutui sta facendo lievitare in forma vertiginosa le espropriazioni immobiliari. A questo punto, complice un alto funzionario del Ministero della giustizia, di cui non ricordo il nome, perché non ho qui *(RC-SE)*. Si fa una convenzione di impiegati esterni *ad adiuvandum* i giudici delle sezioni delle espropriazioni immobiliari, si cacciano gli

che è espressione di un *pool* di banche che ha lo stesso indirizzo di domiciliazione presso l'ABI di Roma. Quindi, l'ABI ha costituito questa società, mettendo i suoi dipendenti esterni *ad adiuvandum*

È un po' come il solito *cliché* della banca del sangue data in appalto a Dracula. Ebbene, abbiamo presentato un'interrogazione, firmata anche da molti altri senatori,

una delle figure più importanti del nostro giornalismo d'inchiesta, in particolar modo televisivo: la dottoressa Gabanelli.

che riguardano i comportamenti delle banche nel nostro Paese: delle banche italiane, ma anche ed in modo particolare Nella sua straordinaria inchiesta dedicata agli *swap* e ai derivati ha fatto emergere e ha portato all'attenzione di tantissimi italiani un fenomeno che vorrei definire una vera e propria bomba ad orologeria, che prima o poi esploderà: forse, allora, qualcuno di questo Governo se ne accorgerà. Ho

forse farebbe bene ad occuparsi di come le banche siano riuscite a penetrare anche nelle stanze del Ministero e ad "aiutare" alcuni fenomeni particolarmente odiosi di sequestri di case a famiglie e a persone non più in grado di pagarsi la rata del mutuo. Le rate dei mutui in questo Paese sono determinate da un sistema di mercato impazzito e fuori da ogni controllo, e le banche del nostro Paese evidentemente non temono l'azione della CONSOB (che, ahimè, troppe volte si è dimostrata fin troppo manchevole da questo punto di vista, deficitaria oltre misura nei casi Parmalat e Cirio, ad esempio): ancora oggi, non solo la CONSOB, ma nemmeno questo Governo si prende cura di informarsi esattamente sulla situazione e sui possibili rimedi da porre in essere, non per aiutare, ma per difendere il diritto dei risparmiatori a non essere utilizzati come carne da cannone dalle nostre banche e, peggio ancora, dalle banche straniere. non solo rivolgo un appello a quelle parti della sinistra che hanno sinceramente e autenticamente più a cuore i destini degli uomini e delle donne di questo Paese, mi spingo a dire che evidentemente questo Governo è espressione di quelle banche e il caso posto da questo emendamento ne è solo un pallido esempio. Vedremo certo una *performance* migliore di questo Governo quando affronteremo l'emendamento sui derivati e sugli *swap* che, in barba ad ogni regola internazionale, sono stati venduti da chi sapeva di vendere merce avariata a tanti Comuni del nostro Paese. Ciò sta riducendo molti Comuni ed alcune Regioni sull'orlo di un fallimento che avviene sotto gli occhi inconsapevoli di tanti di noi, ma certamente con la complicità di questo Governo.

prima casa. Si tratta di una scelta di particolare significato, soprattutto se si pensa - signor Presidente, forse questo non è sufficientemente noto - che quella detrazione è ferma nella sua entità, nella cifra che la determina, da più di dieci anni. Abbiamo attraversato questo lungo periodo sempre lasciando ferma quella detrazione, adesso, sarà anche poco, ma portare in aumento la detrazione

(l'*iter* della finanziaria non è terminato e credo che un impegno politico in questo senso la maggioranza lo potrebbe e lo dovrebbe prendere): non approvare un emendamento come quello al nostro esame, certamente ha una portata finanziaria al di sopra delle possibilità che a questo punto dell'esame della legge finanziaria ci sono, ma intervenire - magari nella lettura della Camera invece di quella del Senato

È chiaro che l'operazione presenta un onere dal punto di vista delle banche; potrebbe esserci un intervento legislativo volto a concorrere a creare le condizioni perché questa diffusa trasformazione dei mutui a tasso variabile in mutui a tasso fisso possa avvenire, possa avvenire, senza criminalizzare nessuno, nemmeno le banche, ma anche riconoscendo che c'è un problema molto serio che si è aperto con la crisi dei mutui *subprime* e bisogna in qualche misura farcene carico. Un primo passo lo abbiamo fatto, un secondo a mio parere si potrebbe fare; l'entità dal passo che ci propone l'emendamento è troppo grande e

abbiamo costituito un movimento politico che, rispetto alle valutazioni e all'analisi della sinistra storica, introduce un elemento dirimente nelle questioni di questi anni. Sono infatti venti anni che il costo del denaro è superiore all'inflazione e ciò ha sottratto enormi risorse finanziarie alle imprese e ai lavoratori. Le banche rappresentano, non solo nel nostro Paese, il vero ostacolo allo sviluppo della democrazia reale con il loro potere sull'informazione, sulla politica e sull'economia, perché il nemico dell'artigiano non è il suo lavoratore e il nemico del lavoratore non è l'artigiano, ma tutti e due hanno la banca che li strozza.

un cittadino che ha contratto un mutuo, ma il profitto della banca rimane inalterato. Bisognerebbe andare nella direzione che indicava il senatore Morando, cioè che quel tasso variabile diventi un tasso fisso e non ci sia tutto il costo a carico del pubblico. l'erba cresce. Ieri è stata occupata la sede dell'ABI da centinaia di cittadini sfrattati perché non riescono più a pagare i mutui.

esprimerò un voto favorevole sull'emendamento 2.50, così come sarei pronto a votare a favore di scelte del Governo che andassero a modificare i tassi da variabili a fissi.

sta acquistando l'Alitalia mettendo ovviamente a rischio il capitale. Vorrei sapere se qualcuno si pone il problema di chi pagherà il rischio dell'acquisto dell'Alitalia; se lo pagheranno le varie persone che hanno contratto il mutuo, le cui case saranno sotto sequestro, o se lo pagherà Pantalone. Mi sembra che nello statuto e nella ragione sociale delle banche non vi sia fare industria.

dall'imposta lorda del contribuente si detrae un importo pari al 27 per cento degli oneri sostenuti a seguito del pagamento degli interessi passivi. Si tratta di una pura e semplice detrazione di imposta di una quota degli interessi passivi.

carico allo Stato di dare un po' ai contribuenti per pagare quei tassi di interesse. Per tale motivo, esprimerò decisamente un voto contrario sull'emendamento 2.50 ed invito gli altri colleghi a non cadere nella trappola che è stata qui identificata.

A questo punto anche le parole del presidente Morando assumono un'altra valenza e non sembrano essere così suggestive di un comportamento virtuoso come invece apparirebbero. Dichiaro il

Il presidente Morando ha ricordato che il Governo e la maggioranza hanno proposto di aumentare di 300 euro

un'entità ridicola rispetto all'incremento delle rate che le famiglie stanno subendo. Giustamente il presidente Morando ha sottolineato che questo tetto di circa 3.700 euro era fermo da dieci anni. Ma il presidente Morando sa meglio di noi che un tetto fisso, quando i tassi d'interesse scendono, significa un sostegno maggiore alle famiglie che debbono pagare il mutuo. Quindi è questo, presidente Morando il momento di dimostrare il sostegno agli italiani, perché è questo il momento nel quale i tassi di interesse salgono

rispetto al dato di fatto, emerso più volte in quest'Aula, anche in questa finanziaria (faccio riferimento anche alla misura sull'IRES), che le vostre manovre sono a vantaggio dei grandi gruppi, delle grandi banche e delle finanza e che vi dimenticate delle famiglie normali e dei lavoratori che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Questa è la verità politica che emerge dal vostro comportamento. In conclusione,